L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che in data 7 giugno 2023 è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche» (747). **Disegni il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e del PNRR:* «Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano» Onorevoli colleghi, come è noto, ieri è venuto a mancare il senatore Silvio Berlusconi. La commemorazione ufficiale del senatore avrà luogo nella seduta di martedì 20 giugno, alle ore 15, ma invito oggi l'Assemblea ad osservare un minuto di raccoglimento in suo ricordo.

La Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha stabilito - in relazione ai funerali di Stato del senatore Berlusconi - di non tenere sedute di Assemblea nelle giornate di domani e di giovedì. Le Commissioni lavoreranno regolarmente giovedì 15 e venerdì 16 giugno. La Conferenza dei Capigruppo ha altresì approvato il nuovo calendario dei lavori fino al 29 giugno. L'Assemblea tornerà a riunirsi lunedì 19 giugno, alle ore 16,30, per la discussione generale del decreto-legge sul rafforzamento della capacità delle amministrazioni pubbliche, approvato dalla Camera dei deputati. Le repliche avranno luogo nella seduta di martedì 20 giugno. Poiché il Governo ha preannunciato la posizione della questione di fiducia sul provvedimento, si è stabilito che si passerà direttamente alle dichiarazioni di voto, alle quali seguirà la chiama. Sempre martedì 20, alle ore 15, si terrà la commemorazione del senatore Berlusconi. Il calendario della prossima settimana prevede inoltre la discussione del decreto-legge in materia di inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro. Gli emendamenti ai decreti-legge in calendario dovranno essere presentati entro le ore 19 di venerdì 16 giugno. Giovedì 22 giugno sarà discussa la mozione Boccia, Patuanelli, De Cristofaro e Unterberger sull'attuazione degli impegni previsti dal PNRR. Il calendario della settimana dal 27 al 29 giugno reca la discussione della terza relazione sullo stato di attuazione del PNRR e, nella giornata di mercoledì 28 giugno, le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 29 e 30 giugno 2023. L'ordine del giorno della seduta di mercoledì 28 prevede la consegna del testo delle comunicazioni rese dal Presidente del Consiglio dei ministri alla Camera dei deputati e, alle ore 15,30, la discussione sulle comunicazioni. I tempi sono stati ripartiti tra i Gruppi per complessive tre ore, escluse le dichiarazioni di voto. Giovedì 29 giugno si svolgeranno il sindacato ispettivo e, alle ore 15, il *question time*. Giovedì 22 giugno, alle ore 9, è convocata la Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia per procedere alla propria costituzione.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

recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche (747) previ